Queste sono costrette ad operare in una situazione di assenza di mercato, in ragione degli impedimenti esistenti non solo per le note posizioni dominanti, ma anche per la complessità del mercato elettrico,

- pensando di risolverne la portata attraverso interventi *spot* molto limitati, che confermano la gravità della situazione. Aver previsto che l'operatore dominante debba cedere al mercato uno *stock* di gas

potrebbe costituire un fattore significativo di riduzione dei costi per le nostre aziende e che questo mercato potrà crearsi solo se

avevamo già presentato un emendamento con il quale si conferiva una delega al Governo affinché assumesse la questione nel suo insieme per risolverla in maniera conseguente.

sul terreno dell'energia, come consumatori finali, subiscono la sperequazione di una disciplina fiscale che le penalizza.

il cui effetto sarebbe neutro dal punto di vista dei costi a carico del bilancio dello Stato. Sulla base dell'invarianza di gettito che verrebbe fuori da questa redistribuzione, crediamo che il principio non possa

che lo consenta.

Cercherò di ribadire, nel tempo che mi è stato concesso, le motivazioni per cui avevamo già espresso il nostro dissenso rispetto a tale provvedimento. Innanzitutto, vorrei ricordare - e per questo era stata presentata una questione pregiudiziale nel corso di questa quarta lettura - che stiamo discutendo di un collegato alla manovra

Effettivamente, Presidente, non riesco neanche a sentirmi. PRESIDENTE. Ha ragione, senatrice, io non so che cosa fare, perché tutti gli appelli cadono nel vuoto.

deleghe in bianco al Governo, che sono assolutamente in contrasto con l'articolo 76 della Costituzione. La nostra contrarietà a tale provvedimento, sempre rimanendo nell'alveo della questione pregiudiziale, si basa anche sul tema della mancanza di copertura finanziaria. Vorrei ricordare ancora una volta in questa mia dichiarazione di voto che non è stata un'opinione del Gruppo dell'Italia dei Valori, ma il

gravate da profili di illegittimità, in quanto assolutamente irrispettose dei principi della contabilità pubblica.

questa previsione è stata completamente stravolta e quindi questo fondo potrà essere utilizzato in qualsiasi modo, non essendoci più alcuna indicazione. Con l'emendamento proposto dal Gruppo dell'Italia dei Valori si voleva in qualche modo reindirizzare questo utilizzo, ma purtroppo esso è stato bocciato, come nella precedente lettura del provvedimento. Voglio anche ricordare che l'Italia dei Valori aveva presentato tutta una serie di emendamenti e ordini del giorno che erano finalizzati a un coinvolgimento reale delle popolazioni e degli enti locali nella localizzazione dei siti per le centrali

Mi avvio alla conclusione sottolineando che la proposta di politica energetica che ha fatto il Governo, e che trova l'appoggio della maggioranza di centrodestra,

per ciò che riguarda il tema dello stoccaggio dei rifiuti radioattivi, sia perché l'Italia dei Valori ha un'idea delle politiche energetiche che, mi permetto di dire, è assolutamente antitetica a quella del Governo in quanto è volta all'attuazione e promozione di una strategia nazionale per lo sviluppo di una filiera industriale per la realizzazione di tecnologie per lo sfruttamento di fonti rinnovabili e all'incentivazione della ricerca e della promozione di tecnologie per l'efficienza energetica e l'integrazione di tali tecnologie. quindi, per una politica energetica che guardi sostanzialmente solo al nucleare. L'ultimo tema che volevo toccare è quello dell'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare

Signor Presidente, colleghi, ci troviamo nuovamente in quest'Aula ad esaminare un provvedimento sul quale il Governo e il Parlamento hanno speso, in tutti questi mesi, profondi sforzi per consegnare al Paese un testo normativo che, se pure esplicherà i suoi effetti in tempi medi e lunghi, pone oggi le basi per un nuova ripresa economica. La crisi in atto nel Paese sta mettendo a dura prova il sistema produttivo, impedendo alle piccole e medie imprese di crescere ed essere maggiormente competitive sul mercato. La portata innovativa di questo provvedimento sta nell'aver concentrato in un unico corpo normativo tutte le misure che via via si sono rese necessarie per affrontare, con una strategia necessariamente influenzata dai profondi cambiamenti nel frattempo intervenuti anche sul piano internazionale, le problematiche strutturali che investono importanti settori strategici dell'economia del nostro Paese. infatti, che è trascorso molto tempo da quando abbiamo iniziato ad occuparci del provvedimento in votazione, ma alla fine questo periodo si è rilevato fondamentale, in quanto ci ha dato l'opportunità di intervenire in modo più consapevole su questioni importanti. Il percorso parlamentare ha permesso, quindi, di ampliare e approfondire le materie trattate, anche se ciò è avvenuto in maniera non sempre lineare e coerente. In particolare, siamo convinti che il Governo debba riprendere e migliorare, ad esempio, la disciplina che regola la distribuzione del gas naturale. Su questo argomento vorrei spendere qualche minuto per ricordare il fatto, grave, accaduto in quest'Aula durante l'esame del provvedimento in prima lettura. L'ex articolo 16*-ter* intendeva sottrarre dalla disciplina generale dei servizi pubblici locali, introdotta dall'articolo 23*-bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, il settore del gas, facendo prevalere quindi sul citato articolo 23*-bis* la normativa di settore. In quell'occasione, il Senato, per salvaguardare le competenze degli enti locali in ordine alla definizione degli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per la distribuzione del gas, ha respinto l'articolo. Nella ripresa della discussione, dopo essere stati coinvolti in un dibattito lunghissimo e, evidentemente, presi sulla stanchezza, ci siamo ritrovati a votare un emendamento proposto dal senatore Lannutti, con parere favorevole del relatore e del Governo, che di fatto ripristina il testo dell'articolo 16*-ter*, precedentemente soppresso dall'Aula. È evidente la contraddizione che emerge dai comportamenti assunti dall'Assemblea. Colgo quindi l'occasione per invitare tutti ad una maggior serietà sul lavoro che siamo di volta in volta chiamati a svolgere. Al di là di questo, il risultato rimane in generale positivo. Al provvedimento va riconosciuto il merito di aver fornito risposte concrete al tessuto delle piccole e medie imprese, ma anche di aver spinto il Paese verso scelte che, soprattutto in campo energetico, si rileveranno fondamentali nel contribuire al benessere dei cittadini e restituire all'intero sistema nuove prospettive di crescita. Sono stati affrontati in modo innovativo molti aspetti importanti che interessano le realtà dei nostri territori e tra questi sono certamente fondamentali per il Nord ed in generale per il Paese le misure adottate per lo sviluppo dei distretti produttivi, la riorganizzazione delle attività di impresa attraverso la creazione di sistemi di rete, la promozione dei prodotti *made in Italy* sul mercato interno ed internazionale e il sostegno alla ricerca. Abbiamo messo mano al rilancio del settore energetico in particolare abbiamo posato la prima pietra per il ritorno del Paese all'energia nucleare che potrà garantire, insieme allo sfruttamento congiunto di tutte le fonti energetiche disponibili, una drastica riduzione dei costi dell'energia a beneficio di imprese e famiglie. Vorrei al riguardo sottolineare che se non operiamo oggi questo tipo di scelte, facendo riferimento alle migliori tecnologie attualmente disponibili in campo nucleare, non potremo domani arrivare ad essere competitivi con quei Paesi che già utilizzano tale fonte di energia. Il Paese si aspetta, quindi, risposte ed è arrivato il momento di fornirgliele per non perdere credibilità di fronte ai cittadini che ogni giorno ci interrogano sul nostro operato. È per tali ragioni che la Lega Nord esprimerà un voto favorevole sul provvedimento.

Non possiamo nasconderci che questo provvedimento, ampiamente discusso sia al Senato che alla Camera, è andato crescendo, anche al di là della sua portata originaria e dei suoi obiettivi:

aspetto che vorrei sottolineare quindi è che, mentre vi sono delle parti del provvedimento che abbiamo contribuito a modificare e sulle quali certamente non vi poteva che essere una condivisione generale (faccio l'esempio delle parti che istituiscono e formalizzano le reti di imprese, o gli interventi a proposito della contraffazione e del contrasto all'alterazione dei prodotti italiani), nel complesso devo dire però che il provvedimento è un'occasione persa per avere una politica industriale del nostro Paese.

sul versante dell'offerta, che invece pare essere l'esercizio migliore di tutti coloro che non intendono affrontare i temi della domanda (e questo provvedimento era un'occasione in tal senso), non si mette in campo una strategia di politica industriale, anzi si rinuncia esplicitamente ad essa. Ma che cos'è la politica industriale? che cos'è la politica industriale? È quella parte della politica economica che si occupa delle imprese, della loro organizzazione, della loro economia e della loro competitività: è quella parte della politica economica che dovrebbe consentire una crescita della competitività del nostro Paese.

sono già stati trasferiti a provvedimenti come la rottamazione ed altri, e sono stati sottratti al sistema generale delle imprese. Non vi sono risorse per le imprese e per la ripresa della loro competitività. Non siamo di fronte ad un provvedimento che guarda alla competitività del Paese neanche quando dice di introdurre il tema di una riforma energetica e dell'energia nucleare.

No, non è una politica industriale comprare da un altro Paese delle centrali nucleari, dare loro dei quattrini, non avere poi i siti dove collocarle, non fare una politica ambientale, né una politica che abbia ricadute sul sistema industriale. di cose diverse. Una politica industriale che guarda al nucleare dovrebbe essere una politica che pensa prima di tutto ad un nucleare italiano e alle potenzialità che dovrebbe avere il sistema imprenditoriale italiano. di un'occasione mancata anche per riaffermare princìpi liberali e di concorrenza dei mercati. Tutte le volte che vi era un provvedimento in campo che dava più forza ai consumatori nei confronti dei monopolisti, il Governo ha scelto i monopolisti: è il caso della *class action*, è il caso della riduzione al silenzio del consumatore nei confronti delle assicurazioni, che vengono riportate ai loro contratti pluriennali, che invece erano stati vietati nella legislazione precedente. Tutte le volte che c'è un monopolista in campo, in questo provvedimento lo ritroviamo come il protagonista privilegiato. Tutte le volte che c'è un concorrente lo ritroviamo messo nell'angolo da una concorrenza che viene negata, da un mercato che non viene dispiegato. Tutte le volte che c'è un consumatore, sentiamo che questo consumatore deve ridurre le sue pretese perché si debbono affermare invece le mani libere di un mercato senza regole, le mani libere di monopolisti senza scrupoli, ma anche le mani libere di un Governo

che dovrebbe controllare, e in qualche modo stimolare, gli effetti generali della politica nucleare - per riprendere quest'Agenzia alle proprie dipendenze: mani libere, quindi, verso una politica senza controllo.

quelle che hanno tolto di mezzo la *class action* - o almeno ne hanno impedito l'attuazione - oppure le disposizioni sul trasporto ferroviario e sul trasporto pubblico locale, sulla rivalutazione contabile dei titoli. In buona sostanza, l'originario disegno di legge è diventato un provvedimento *omnibus* nel quale si è ricompreso di tutto, ma questo "tutto" corrisponde ad una concezione non liberale, non competitiva, non aperta del mercato, ma a quella di un mercato vincolato e in qualche modo politicamente guidato, che non consente al sistema delle imprese italiane di crescere sul piano della competitività.

Onorevole Presidente, colleghe e colleghi, signor ministro Scajola, finalmente, dopo tanto lavoro, stiamo per approvare un testo di importanza fondamentale, mi permetterei di dire storica, poiché rappresenta una svolta radicale in tema di politica energetica per il nostro Paese e un deciso scatto in avanti per ciò che riguarda lo sviluppo delle imprese. Il testo che torna dalla Camera dei deputati non presenta sostanziali stravolgimenti dei capisaldi della riforma per la crescita e lo sviluppo del sistema economico-industriale fissati durante l'esame in Commissione industria, prima, e nell'Aula del Senato, poi, ma recepisce alcune mirate osservazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, a dimostrazione della collaborazione proficua dei vari Ministeri interessati e della convinta maggioranza parlamentare che appoggia l'attuale Esecutivo. Il disegno di legge che andiamo ad approvare può essere sinteticamente riassunto in tre grandi tematiche socio-economiche: riordino del sistema energetico nazionale, con particolare riguardo al tema del nucleare, incentivi all'aggregazione tra imprese e difesa dei diritti dei consumatori. Temi di preminente interesse nazionale che per questo vanno con forza sostenuti. Sessanta miliardi di euro all'anno, quattro punti percentuali di PIL: tanto è il costo della bolletta energetica che grava sulle famiglie italiane, ma soprattutto sui bilanci del sistema produttivo nazionale.

Dipendere dal punto di vista energetico quasi interamente da altri Paesi condiziona non poco, da un punto di vista geopolitico, l'azione strategica dello sviluppo economico del Paese, che non può sottostare ai *desiderata* altrui. In questo senso vorrei ricordare l'opera intelligente e concreta svolta dal ministro Scajola in questo anno durante il quale ha percorso in lungo e in largo i sistemi Paese di altri Stati per rafforzare la nostra indipendenza dal punto di vista energetico. La conclusione è una sola: diversificare quanto più possibile il fabbisogno energetico e puntare decisi alla produzione di energia derivata dal nucleare, cercando di colmare quel *gap* tecnico che, in modo miope e colpevole, ci ha differenziato negli ultimi trent'anni dagli altri Paesi europei. Il processo di avvicinamento alla produzione di energia da nucleare avverrà sotto comuni denominatori: sicurezza, rispetto per l'ambiente e garanzia per la salute dei cittadini. Priorità, queste, che l'attuale Esecutivo ha ben presenti, ma che non possono prescindere dalla necessaria azione di sviluppo che obbligatoriamente deve accompagnare l'attuale fase di rilancio del sistema imprenditoriale. Non liberismo senza regole, come qualche maligno tenta di insinuare, ma la consapevolezza che senza ricchezza e ripresa dell'economia vengono messi in dubbio i valori fondamentali dello Stato sociale. Il testo che andiamo ora a licenziare va proprio in questo senso, nella certezza che lo sviluppo del Paese viaggia di pari passo con l'ammodernamento della propria rete energetica. Nucleare sì, ma con tutti i presupposti di trasparenza e sicurezza necessari. la previsione di una delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo, recanti criteri per la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare,

altresì - come noto - la costituzione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, leggermente modificata nel ritorno dalla Camera, che avrà le funzioni e i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza delle attività concernenti gli impieghi pacifici dell'energia nucleare.

attraverso la creazione di un apposito Albo delle imprese cooperative, nonché una serie di misure aventi come finalità quella di semplificare le procedure burocratiche tese al rilascio di titoli autorizzativi o concessori da parte della pubblica amministrazione. Il provvedimento reca poi importanti misure in ambito di difesa dei diritti dei consumatori. È di questi giorni la polemica aperta dal ministro Scajola rispetto alle dichiarazioni rilasciate da alcuni settori produttivi per quanto concerne il prezzo della benzina. Basterebbe ricordare le dichiarazioni del Ministro in occasione della riunione dell'Unione petrolifera: qualcuno

abbiamo svolto un'indagine conoscitiva sui prezzi dei prodotti petroliferi, di cui sono particolarmente fiero per il contributo fornito in termini di contenimento dei prezzi alla pompa, contributo che ha dato la possibilità al Ministro di sostenere questa polemica. Sempre in tema di sicurezza e a difesa della qualità del servizio reso ai cittadini, si segnalano importanti disposizioni recate dal testo in esame in tema dei requisiti necessari per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale. Si dispone, infatti, che per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri aventi origine e destinazione nel territorio nazionale, per i quali sia necessario l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale, le imprese ferroviarie debbano essere in possesso di apposita licenza

delle imprese, dei lavoratori, ma soprattutto, mi sia consentito, dello spirito unanime della maggioranza e del Governo, che su un tema così delicato hanno dimostrato unità di intenti, chiarezza di idee e volontà di risultato.

Un grazie ai colleghi tutti che in Aula hanno voluto con concretezza dare il loro contributo. Il Governo, e il ministro Scajola in particolare, ha saputo capire il nuovo che c'è nel Paese ed in Europa, così come il G8 di queste ore ci sta dimostrando, con apprezzamenti estremamente positivi e lusinghieri che sono sulla stampa, su ogni giornale, italiano o straniero.

alla sfida dell'innovazione per essere al passo dei tempi con positiva determinazione e volontà di fare, per dare a questo nostro Paese sempre di più la possibilità di concorrere, a livello nazionale ed europeo, alla grande sfida che si è aperta.

Signor Presidente, visto e considerato che è stato deciso mesi fa di far svolgere gli interventi sull'ordine dei lavori a fine seduta e oggi addirittura si sospende la seduta per far uscire tutti, magari anche i membri del Governo ai quali ci si voleva appellare per ricordare alcune interrogazioni parlamentari, io non so che dire: eravamo la serie B e adesso siamo diventati addirittura la serie C. Non si riesce a capire come mai, visto e considerato che poi tutti restano in Aula a parlare di questioni che vanno sicuramente a toccare i nodi fondamentali del nostro lavoro parlamentare, si debba addirittura sospendere per cinque minuti i lavori prima di iniziare questa fase. Naturalmente non mi ero iscritto a parlare per questo, ma

Alla vigilia del G8 il presidente cinese Hu Jintao è tornato di corsa a casa propria perché la situazione nello Xinjiang, nel Turkestan orientale, è peggiorata.

Da ieri i deputati Mecacci, Zamparutti, Bernardini, Farina Coscioni, Turco, Giachetti ed io siamo in sciopero della fame per chiedere al G8 che

solo nelle zone dove si riesce a percepire la violenza degli uiguri contro i cinesi e non la repressione dei cinesi contro gli uiguri e che si avvii un cammino di riconciliazione fatto di proposte politiche e non soltanto di risposte militari

si è finalmente ed opportunamente aperto un dibattito sui cittadini non comunitari, che sappiamo tutti essere presenti nel nostro Paese, per i quali - come tutti sappiamo - i loro datori di lavoro

dallo Stato italiano a lavorare in clandestinità e in nero.

Presidente, il G8 è iniziato ufficialmente ieri ma c'è una parte di Roma che da qualche giorno è vietata al transito pedonale e veicolare. Questa parte di Roma ha un nome: si chiama via del Plebiscito. Sono quattro giorni che sul tratto di via del Plebiscito dove casualmente vi è la residenza privata di un noto personaggio delle istituzioni non si può transitare né a piedi né in macchina.

sul tratto di via del Plebiscito tra piazza Venezia e piazza del Gesù è una cosa che grida vendetta al cospetto di Dio. È una cosa vergognosa, signor Presidente, anche considerando tutti gli attestati di riconoscibilità personale o di *status*

mi è stato risposto che dovevo girare da un'altra parte per motivi di sicurezza pubblica. Io trovo che questa sia una cosa vergognosa, signor Presidente, e le chiedo la cortesia, nelle forme e nelle modalità che riterrà più opportune, di far pervenire la protesta formale del sottoscritto, se è l'unico, e degli altri che la volessero condividere al sindaco di Roma, al prefetto, nella sua qualità di responsabile del Comitato provinciale per

uomo arrestato e condannato fosse in libertà e fosse il capo di una banda di malfattori che, il giorno 6 di questo mese, ha assaltato un portavalori nella Regione Lazio.

Signor Presidente, anch'io vorrei sollecitare il Governo a rispondere alle numerose interrogazioni parlamentari presentate dal sottoscritto in merito a quella che sta diventando una vera e propria telenovela, ossia la vicenda Quell'azione di classe, che doveva entrare in vigore - ce lo ricordiamo tutti - il 1º luglio 2008, è stata rinviata al 1º gennaio 2009, poi al 1º luglio 2009 e ancora a data a data da destinarsi - cioè alle calende greche, come si suol dire - non si sa bene perché. Voglio solo far notare a lei, signor Presidente, ed anche ai colleghi che ci ascoltano, che la mancanza di queste

con la rinegoziazione dei derivati il Comune di Milano, come risulta dalle intercettazioni telefoniche depositate alla procura di Milano da parte del pubblico ministero Alfredo Robledo. Signor Presidente, questa è davvero una telenovela,

di tantissime altre frodi a danno delle famiglie, dei più anziani e soprattutto delle persone più indifese. E questo Governo, che si vanta di essere paladino del mercato,

sarà rappresentato in Consiglio di Presidenza. Ma noi non vogliamo entrare dalla porta di servizio, caro Presidente: noi vogliamo entrare come si doveva entrare un anno fa, cioè dalla porta principale con le deleghe giuste, che potevano essere quelle designate il primo giorno del primo anno di questa legislatura. Ad oggi continua ancora l'umiliazione

può dire o esprimere parere contrario; non possiamo farlo in un organo da cui ci hanno volutamente escluso un anno fa. Continuiamo a non capire e continuiamo a denunciare questo fatto. Non accettiamo parole di conforto e spero che non ce ne siano dopo il mio intervento, perché queste parole ad oggi si sono rivelate un'autentica

che il quarto Gruppo dell'Aula del Senato non sia presente in Consiglio di Presidenza è qualcosa che non va bene, perché